L'esercizio delle funzioni costituzionali assegnate alle Camere presuppone la loro capacità di assumere correttamente le decisioni. In pratica, il fenomeno «pianistico» in generale e, in particolare, in relazione a ciò che è accaduto questa mattina in Aula abbisogna di una doverosa riflessione. Sappiamo che l'articolo 64 della Costituzione non ammette il voto per delega, il voto è personale quando ci sono delle irregolarità nell'esercizio del voto le votazioni vanno annullate ai sensi dell'articolo 118, comma 1, del Regolamento. Questa mattina un Ministro della Repubblica dai banchi del Governo ci ha dimostrato di essere un bravo pianista. Il ministro Bondi che, non vergognandosi di quello che ha fatto durante tutta la gestione*...(Proteste

perché, se è vero che il Regolamento usa l'avverbio "immediatamente" (immediatamente, ancorché la Presidenza ne avesse contezza: la Presidenza, come al solito, era evidentemente un po' distratta) tutti i siti *web* d'Italia, di tutti i principali di tutti i principali quotidiani italiani mostrano un comportamento vergognoso come quello che la maggioranza sta avendo in questo frangente. Quindi, chiedo alla Presidenza non solo l'annullamento di un imbroglio, che il *web* sta mostrando ormai in Italia, e oltre, di un Ministro della Repubblica che bara al momento del voto...

Questa è la prima richiesta che noi facciamo. La seconda richiesta, che facciamo in via subordinata, è che venga convocata con urgenza sul punto la Giunta per il Regolamento. Regolamento. Concludiamo chiedendo, prima di una sfiducia votata dal Parlamento, uno scatto d'orgoglio, se ancora ne è rimasto al ministro Bondi: si dimetta una buona volta!

Presidente, non intendo in alcun modo alzare i toni del dibattito, ma vorrei semplicemente consigliare al senatore Belisario - che evidentemente

della seduta di questa mattina. È accaduto che un senatore della sinistra, dell'opposizione, abbia interloquito con il presidente di turno Nania,

ha chiesto al Presidente, in maniera anche evidente ed accesa, di rivedere quella citazione, tra virgolette, inopportuna.

ed evidentemente rimetteva, non una denuncia, ma una semplice citazione. Questo è il modo con cui ci si comporta tra colleghi e tra gentiluomini in un'Aula come quella del Senato. PdL)*. In una situazione del genere, il collega Belisario doveva almeno avere la precauzione di chiedere al ministro Sacconi, che è qui presente,

conosciamo le prassi in quest'Aula - e che tale denuncia ha un peso se il ministro Sacconi fosse stato assente; ne ha completamente un altro, e diventa semplicemente una strumentalizzazione, nel caso in cui il ministro Sacconi

sul conto il crollo di alcuni edifici di Pompei; addirittura si è affermato che ha violato la Costituzione. Non si capisce perché, quando è caduto il tetto della cattedrale di Noto,

come è noto, frequento quest'Aula con la stessa assiduità con cui lo fa il collega Quagliariello. Noi abbiamo posto un problema che è consacrato in immagini televisive... che tutti gli italiani stanno vedendo sul *web.* Il ministro Bondi, anziché venire in Aula e dire, come spesso mi capita, «ho sbagliato anche questa mattina» si trincera dietro strane giustificazioni addotte dal collega Quagliariello...

Noi abbiamo posto un problema reale, non è fantasia. Le giustificazioni non sono ammesse sul fenomeno

Ignazio Marino era presente in Aula e ha chiesto espressamente al senatore Carofiglio di votare per suo conto per suo conto in sua presenza. Se lo stesso è accaduto al ministro Sacconi ci sarebbe piaciuto sentirlo dire e raccontare dallo stesso Ministro e non dal difensore d'ufficio. Detto questo,

mi dispiace dover fare una citazione di ciò che io chiesi al presidente Schifani - richiamando il fatto che in questa legislatura era stata introdotta un'innovazione importante (mi ascolti signor l'innovazione importante è che sono stati assegnati i posti, cosa che non era prevista nelle passate legislature. In ragione di tale innovazione, chiesi al Presidente Schifani, per evitare questo fenomeno sempre più ricorrente, di adottare un sistema semplice, cioè di disporre che gli assistenti parlamentari, e non i senatori Segretari (che hanno una funzione di controllo),

soppressione del primo e del terzo periodo del comma 8 dell'articolo 5,

sulla sabbia, fatto di 173 norme, 500 regolamenti e quant'altro, si regge persino su una sorta di pagherò,

questo tipo di testo. Faccio appello anche al Presidente della Commissione e all'ex relatore, senatore Asciutti: non lo possiamo permettere: è gravissimo fare questi errori, anche in termini meramente giuridici. comma 8 è scritto molto male, è incomprensibile, è un cattivo esempio di italiano e bisogna provvedere a modificarlo, bisogna avere il coraggio di riconoscere i propri errori, come penso poc'anzi avrebbe potuto fare anche il ministro Bondi.

faccia togliere le schede dove non ci sono senatori, in adempimento di un obbligo e di una decisione assunta.

stiamo seguendo delle procedure che verosimilmente sfioreranno il ridicolo. Parto da un presupposto: le schede, per poter essere inserite, debbono essere ritirate dal senatore all'interno dell'Aula. Quindi si dà per scontato che il senatore è venuto, ha ritirato la scheda e l'ha inserita. Può accadere che il senatore si debba spostare per una serie di motivi, compreso il colloquio con un altro collega in riferimento agli argomenti che si stanno discutendo, o comunque per quelle interlocuzioni ordinarie che ci sono in un'Aula parlamentare *(Applausi dal Gruppo PdL)*, e non in un recinto che viene picchettato. Può accadere che vi siano problematiche di carattere fisiologico, può accadere che si esca per altri motivi: e, nel momento in cui si rientra, bisogna rifare

Senatore Tofani, la ringrazio per il suo contributo, però io rinnovo il mio invito. Se il senatore non è seduto al proprio posto, perlomeno tolga la scheda e la lasci sul banco, così evitiamo di continuare a discutere su chi deve votare e per chi si deve votare. ***Votazione nominale con

Da un lato si elimina il riferimento alla legge n. 230 del 2005 e dall'altro si inserisce per intero il testo della legge in questione

per vedere come si stia tacendo su delle autentiche oscenità giuridiche e formali che la Camera ha apportato. Per questa ragione chiediamo di ripristinare integralmente il testo che avevamo approvato in prima lettura.

alla Camera hanno combinato un pasticcio evidente sul testo.

della legge 4 novembre 2005, n. 230. Con questo comma si provvede ad una riscrittura della norma. Il successivo comma 5, di cui noi chiediamo la soppressione, modifica lo stesso comma

del vecchio articolo 1 della legge n. 230 del 2005. Sta di fatto, però, che questo obiettivo viene conseguito con due testi,

Quindi, l'articolo 1 della legge n. 230 del 2005 una volta viene riscritto, un'altra volta viene modificato e un'altra volta ancora abrogato. Mettetevi d'accordo voi: tutte e tre le cose sicuramente non si possono fare. Noi avremmo una soluzione da suggerire, ma non ci permettiamo Credo che la Presidenza sia assolutamente in grado di valutare e di decidere. Ciò che è certo è che questo testo di legge, così come scritto, non può rimanere: questo è sicuro. Il suggerimento immeditato è quello di abrogare il comma 5, che è l'oggetto dell'emendamento. Su questo aspetto, signor Presidente, potendo esso costituire un precedente molto serio, la prego di assumere una decisione che sia chiara.

è già successo con altri Governi. In questo caso, il Governo si impegna a risolvere il problema in sede di provvedimento

un refuso o una parola al posto di un'altra. In questo caso ci sono tre commi che si riferiscono allo stesso articolo proponendo soluzioni tra loro diverse.

la Presidenza si limita a precisare quanto segue. Sebbene sia sostenibile che il testo dell'articolo 6, come modificato dall'altro ramo del Parlamento, presenti una potenziale contraddizione formale con l'abrogazione prevista all'articolo 29, comma 11, del medesimo disegno di legge, non pare alla Presidenza che questa si risolva in un rischio di violazione del divieto di porre in votazione proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Senato. Infatti, dalla lettura dell'intero articolo 6 e dall'interpretazione sistematica del testo del disegno di legge al nostro esame, appare chiara ed intellegibile la disciplina espressamente recata dall'articolo 6, comma 4. Comunque si voglia intendere l'apparente contrasto tra l'abrogazione prevista all'articolo 29 e la modifica della stessa norma recata dall'articolo 6, comma 5, il citato comma 4 riscrive per intero la disciplina dell'attribuzione del titolo di professore aggregato. La Presidenza, naturalmente, non entra nel merito della scelta risultante dalle votazioni - effettuate dalla Camera dei deputati sul testo originariamente deliberato da questa Assemblea - ma si limita a evidenziare che la riscrittura della norma al citato comma 4, al di là dell'abrogazione espressa di cui all'articolo 29, opera una abrogazione implicita dell'articolo 1, della legge n. 230 del 2005. E ciò vale a scongiurare ogni rischio che questa Assemblea incorra in deliberazioni contraddittorie. Rimane impregiudicata, naturalmente, la facoltà da parte del Governo di proporre e sostenere, in futuro, eventuali interventi normativi volti a tornare sull'argomento, anche al fine di rendere la disciplina ancora più chiara e lineare e migliorare la qualità normativa di questa parte del testo della riforma.

Presidente, la soluzione che la Presidenza ha ritenuto di sottoporre all'Assemblea io la giudicherei fantasiosa. fantasiosa. Adopero questo aggettivo per essere il più possibile rispettosa della Presidenza e degli Uffici. Noi stiamo sostenendo in quest'Aula,

al comma 5 dello stesso articolo, torniamo ad intervenire sullo stesso comma 11, apportando le stesse modifiche che con il comma precedente abbiamo apportato riscrivendo l'articolo; successivamente, all'articolo 29, abroghiamo lo stesso Ora, francamente non ho idea di come la Presidenza possa ritenere di risolvere tale questione perché, nel momento in cui la legge verrà approvata, e successivamente promulgata, avremo dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230 che, letto sistematicamente, non è più quello originario, bensì quello modificato, e lì potremo scegliere se nella formulazione dell'un comma o dell'altro, e in quanto tale abrogato, mentre a questo punto è possibile che sopravviva

Ma neanche sotto il profilo della regolarità del procedimento legislativo questa soluzione funziona. Non soltanto nel momento in cui la legge verrà approvata e promulgata, ma neanche sotto il profilo del procedimento amministrativo potrà mai funzionare. La verità è che per non cambiare una virgola virgola di un testo che noi non condividiamo - ma questo è un altro paio di maniche - ma che è un pasticcio assoluto, voi perseverate e create precedenti che sono contro la migliore tradizione legislativa, o meglio l'ordinaria tradizione legislativa, di qualunque Parlamento del mondo.

Signora Presidente, gli argomenti dei colleghi del Partito Democratico appaiono del tutto inoppugnabili. La conseguenza che nascerebbe dal proseguire con questo sistema è fotografabile con un'espressione della massima semplicità. Si stabilisce un pericoloso precedente per cui, nella confezione di una legge, un articolo, o un comma, può essere uno e trino:

dietro richiesta dell'opposizione, che lamentava l'anomalia di quel caos che aveva dato luogo a quelle votazioni sulle quali la Presidenza era andata avanti nonostante le richieste di sospensione d'Aula, avevo detto ai Capigruppo di maggioranza e di opposizione che la mia intenzione era quella di di procedere alla rinnovazione di quelle votazioni, perché non si era verificata la rispondenza dello stato di conoscenza tra il senatore e quello che si stava votando. Questo avevo detto, e ne sono testimoni sia i Capigruppo di maggioranza che di opposizione,

aveva deciso, su richiesta dell'opposizione, di ripetere quelle votazioni che erano state effettuate in una fase di caos. Quindi, la Presidenza ha agito in maniera del tutto trasparente e in perfetta buona fede. Buona fede che consente, a questa Presidenza, di rinnovare e confermare questa sua decisione, coè di ripetere quelle votazioni. Sovviene in tal senso anche l'articolo 118, comma 1, del Regolamento, che prevede che prevede che: «In ogni caso di irregolarità delle votazioni, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullarle e disporne l'immediata rinnovazione, con o senza procedimento elettronico». Io cito precedenti Io cito precedenti di questa Presidenza che, addirittura, ha fatto rinnovare, su richiesta dell'opposizione, votazioni elettroniche (ed è la storia che lo dice).

la seduta era diversa e si sarebbe dovuto rinnovare, o procedere alla rinnovata votazione, in una seduta diversa da quella in cui si era effettuata la votazione oggetto di contestazione. nel corso della stessa seduta e mi sento quindi, in piena coscienza, di poter ribadire e affermare quanto già avevo deciso prima ancora di sapere dell'esistenza del problema, cioè che queste votazioni sono state effettuate in un momento di irregolarità, perché è chiaro che, in un momento in cui vi è caos in Aula

possano avere a mente un problema. Noi stiamo vivendo un momento delicato, anche sotto il profilo delle tensioni esterne. Pertanto, io sarei felice se da questa Aula, nel rispetto delle posizioni, venisse intrapreso un dibattito che rispetti i termini della dialettica e non della conflittualità, perché ne abbiamo già parecchia all'esterno.

Signor Presidente, noi sappiamo bene, perché conosciamo il Regolamento, quali sono le sue facoltà; però credo che, proprio per un esercizio pienamente responsabile della nostra presenza in quest'Aula e per il fatto che l'esercizio responsabile è anche quello, forse soprattutto quello, di non lasciare angoli bui nella discussione tra maggioranza, opposizione e Governo, sia necessario fare alcune considerazioni. Tutti ricordano come è cominciata questa discussione in Aula. È sorta da un'obiezione sollevata dal collega Legnini, che ha osservato - in maniera corretta e del tutto inoppugnabile, peraltro perché testuale, come del resto ammesso dalla stessa ministro Gelmini poc'anzi

comma 11 dell'articolo 1 della cosiddetta legge Moratti, un secondo comma dello stesso articolo prevedeva una riformulazione per il mezzo di inserzioni nel testo originario,

valgono a fare del testo in via di approvazione non soltanto un testo sul quale il Senato si esprime in maniera intelligibile, ma un testo con una sua congruità. Esiste nell'altro ramo del Parlamento un Comitato per la legislazione, nato esattamente per questa ragione, e sono riconosciute responsabilità anche nel Governo Governo affinché ciascun testo abbia una sua compiutezza e sia in grado di inserirsi armonicamente nell'ordinamento, perché la leggibilità della regola vale soltanto ai fini della sua applicazione, ma anche a quelli della sua piena conoscibilità da chi è chiamato ad osservarla. Se dunque siamo qui nel potere di fare le leggi, abbiamo però il dovere di farle intelligibili, conoscibili, razionali, logiche.

un testo così interpretativo, talmente interpretativo, da doversi fare ricorso al criterio dell'interpretazione sistematica per giustificare che, nello stesso testo, vi fossero norme così in contraddizione palese fra loro. Tutti i colleghi ricorderanno che a quel punto io sono intervenuta contestando da una parte il procedimento legislativo, così come si sarebbe svolto sulla base dello dello *speech* letto dalla presidente Mauro e che io ritengo assolutamente non adeguato al momento del farsi della legge e delle votazioni, dall'altra parte chiedendo che, esattamente per la regolarità del procedimento legislativo e per adottare il principio che ci assistesse nel prosieguo dell'esame dal testo, così impervio per le ragioni anzidette, venisse convocata la Giunta per il Regolamento. A questo punto, Presidente, è successo ciò che non dovrebbe accadere, e cioè che, a questa protesta dell'opposizione, che non riguardava il merito, il contenuto del testo, ma era una protesta - peraltro civile, penso - orientata a garantire la regolarità del procedimento legislativo e l'osservanza del Regolamento, è stata data una risposta - mi perdoni se adopero questo aggettivo - prepotente

che non riusciva ad ottemperare a nessuna delle osservazioni che avevamo fatto, si è continuato nel tumulto a porre in votazione gli emendamenti, a riprova della presenza in quest'Aula di una maggioranza che è in grado di fare tutto da sé, ignorando le richieste, le proposte e anche i rilievi dell'opposizione.

con una forza e una prepotenza alla quale non eravamo neanche preparati, si è continuato a porre in votazione gli emendamenti.

È vero, lo sanno anche i colleghi che mi hanno visto nell'emiciclo fare un mestiere che normalmente svolgono soggetti di altra prestanza fisica, davanti alle discoteche.

frattempo, Presidente, è successo un altro fatto. Non solo la presidente Mauro ha continuato - e continua tuttora - ad insistere circa la regolarità della propria dichiarazione in ordine all'esito delle votazioni, ma il mondo

Ciò nonostante, si è continuato, perché era una prova di forza. Ebbene, quest'Aula, su tali questioni, su questo tema, in questo momento non può essere chiamata ad una prova di forza. Voi ci chiedete di essere responsabili: noi chiediamo a voi e al Governo di essere responsabili almeno quanto lo siamo noi.

questo testo al termine della votazione che compiremo nella giornata di domani, poiché contiene norme di cui l'una elide l'altra, l'una costruisce, l'altra modifica e l'altra ancora cancella.

sette imposte all'Aula mentre l'Aula è in subbuglio! Questa è la nostra posizione. Le avevamo promesso che avremmo mantenuto nell'esposizione delle nostre buone ragioni un profilo di di chiarezza, ma anche di responsabilità - chiamiamola così -se responsabilità è il pronunciarsi in un'Aula con i modi che si convengono alla Mi augurerei che da parte di tutti gli altri soggetti di questa vicenda di oggi ci fosse lo stesso senso di responsabilità per quello che qui accade e per quello che comunque fuori da qui sta già accadendo. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi ovviamente ci stiamo muovendo nell'ambito del Regolamento, cercando anche di applicare il buon senso al quale lei ha richiamato. Sappiamo che nelle Aule spesso si possono vivere dei momenti di tensione e di clamore, tanto è vero che l'articolo 68 del nostro Regolamento prevede casi di questo tipo: tipo: qualora dovessero sorgere in Aula dei tumulti, il Presidente sospende la seduta abbandonando l'Aula, allontanandosi, e la seduta riprende con il ritorno nell'Aula del Presidente.

È soltanto il Presidente che può decidere se quello che sta accadendo in Aula è a suo giudizio un tumulto, sicché, ai sensi dell'articolo 68, sospende la seduta, oppure ritenere che quello che accade in Aula, pur in in un momento di tensione e di clamore, non configuri l'ipotesi prevista all'articolo 68. La presidente Mauro ha, all'evidenza, liberamente e nell'ambito dei suoi esclusivi poteri, poteri, apprezzato che ciò che accadeva in Aula non era tale da imporre la sospensione della seduta, ossia non ha ritenuto di dovere applicare l'articolo 68 Ad esplicita richiesta di alcuni nostri colleghi che invitavano alla sospensione della seduta, la Presidente ha espressamente affermato che non riteneva di dover interrompere i lavori. Quindi, ha liberamente apprezzato ciò che rientra nell'ambito della sua esclusiva prerogativa. Avendo ciò fatto e avendo ritenuto che i lavori potessero continuare, a qualche collega che diceva "ma noi non sentiamo quali emendamenti si votano" la Presidente Mauro ha specificato che il numero dell'emendamento che andava in votazione era chiaramente percepibile. Queste sono le dichiarazioni registrate.

ha proclamato il voto pronunziando la parola: approvato. In tre occasioni, ai sensi dell'articolo 111 del Regolamento, la Presidente ha proclamato il voto dicendo: non approvato. Sicché, ha dimostrato una totale possibilità di dominio del momento di tensione, diversificando il risultato del voto e proclamandone l'esito: in quattro casi, con la pronunzia di approvato, in tre casi con la pronunzia, di non approvato. Lei ora, signor Presidente, ritiene che si possa applicare l'articolo 118 L'articolo 118 prevede la possibilità dell'annullamento del voto irregolare che deve avvenire immediatamente, questa è una prerogativa che ovviamente appartiene al Presidente nel momento in cui verifica che l'espressione di quel voto sia connotata da irregolarità. Ma questo non è stato fatto dalla presidente Mauro: a distanza di circa due ore lo sta facendo lei, Presidente. E non sta annullando un voto irregolare: sta proponendo l'annullamento in blocco di sette voti.

annullare sette voti, cioè un'intera fase dei lavori d'Aula,

non ha ritenuto che esistessero le condizioni che lei, a distanza di due ore, ritiene ora per allora esistenti. Ma in questo modo noi violiamo anche le prerogative della Presidenza, introduciamo un precedente gravissimo: a distanza di tempo si può annullare un voto perché si può assumere che la percezione di quanto è accaduto in Aula era una percezione che doveva essere confinata nell'ambito del tumulto e non valutabile diversamente da chi in quel momento presiedeva l'Aula. Questo non si può fare. Noi stiamo dicendo che chi presiede l'Aula ha dei poteri limitati, perché ci può essere il Presidente che arriva dopo - che può essere il Presidente del Senato ma anche un Vice Presidente - il quale valuta dopo ciò che era accaduto prima e apprezza dopo ciò che prima non era stato apprezzato. Non è possibile che si faccia una cosa del genere: introdurremmo un criterio veramente discrezionale su materia che per sua natura è discrezionale, signor Presidente. È la sua stessa natura. È l'apprezzamento che dà chi presiede. che tutto ciò che avviene nell'Aula è dominio del Presidente; anche la polizia dell'Aula appartiene al Presidente, che la esercita la esercita attraverso i funzionari, ma è una sua prerogativa. In questo caso, non è stata esercitata; non si introduca introduca l'interpretazione di una percezione che il Presidente del momento non ha avuto facendo proclamazioni differenziate; non si faccia a distanza di due ore ciò che poteva essere fatto due ore prima. Oggi, infatti, introdurremmo una violazione gravissima del Regolamento. I Regolamenti hanno rango costituzionale: sono leggi che appartengono alla nostra Costituzione e non sono liberamente interpretabili o applicabili.

può sospendere la seduta perché c'è tumulto in Aula, è quel Presidente che la può sospendere; se si afferma che il Presidente, e soltanto lui, può proclamare il voto dicendo

la seconda questione riguarda la corretta applicazione dell'articolo 97 del Regolamento in ordine all'ammissibilità di alcuni emendamenti che sarebbero in contrasto con precedenti deliberazioni adottate da quest'Assemblea.

di un errore commesso dalla Presidenza e frutto, cari colleghi della maggioranza, della vostra supponenza in un momento così delicato dal punto di vista politico ed istituzionale per il Paese, nel momento in cui ci troviamo in questa circostanza Io credo sarebbe opportuno che ci diamo tutti una calmata e cerchiamo di capire che anche la tifoseria da stadio in certi momenti - e quindi fare il tifo per la Presidenza di turno - diventa un *boomerang* per quest'Aula e per i fatti che abbiamo davanti.

che la Giunta per il Regolamento deve affrontare. L'affronterà stasera; se fosse stato fatto due ore fa probabilmente non saremmo a questo punto, ma credo che sia corretto ciò che viene chiesto dai colleghi del Partito Democratico. Detto questo, credo che obiettivamente noi dobbiamo cercare, per quello che è nelle nostre possibilità, di coniugare l'esigenza di dare a quest'Aula la possibilità di esprimersi serenamente sugli emendamenti garantendo la corrispondenza tra la volontà dei senatori e la decisione (quindi il voto) assunta sui singoli emendamenti (ciò che non è stato garantito e non per colpa delle opposizioni, ce ne vorrà dare atto) e l'esigenza che il modo di procedere nella votazione sia logico e consequenziale e non porti a deliberazioni che siano in contrasto fra di loro su singoli emendamenti, perché, questo sì, qualora fosse in punto di fatto e di merito vero, sarebbe in contrasto con la norma regolamentare. Ma poiché se aprissimo una discussione su questo punto la concluderemmo fra una settimana, credo sarebbe più opportuno che lei rimetta la questione alla Giunta per il Regolamento e noi si continui ad andare avanti, per quello che è possibile, serenamente con i nostri lavori.

Per fare una breve cronistoria di ciò che è successo e per evitare mistificazioni come quelle che ho sentito negli interventi che mi hanno preceduto, ricordo che la presidente Mauro si è limitata a leggere lo *speech* che le è stato proposto dagli uffici. Una volta letto, lo *speech* diventa la posizione ufficiale della Presidenza del Senato; non è un'opinione personale della vice presidente Mauro, ma diventa una posizione ufficiale della Presidenza del Senato. Dopo la lettura dello *speech*, le opposizioni hanno iniziato ad attaccare, non solo verbalmente, i banchi del Governo e quello della Presidenza. Questo è avvenuto ancor prima che si mettessero ai voti gli emendamenti tanto contestati. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

La dimostrazione è nel fatto, cari colleghi, che una volta sospesa la seduta, tutti i Capigruppo, di maggioranza e di opposizione, hanno convenuto insieme, su richiesta delle opposizioni, di ripetere le votazioni degli emendamenti che erano state fatte in Aula, perché non erano avvenute regolarmente. Questo è stato detto dalla presidente Finocchiaro, dal presidente Belisario e da tutti i Capigruppo dell'opposizione: dobbiamo ripetere le votazioni perché non si sono svolte in un clima sereno, in modo regolare. E tutti abbiamo accettato.

Presidente, in via di estrema sintesi, io credo che il tema sia la cultura delle regole. Non penso si possa non riconoscere che, ad un certo punto del dibattito in Senato, questo principio nella pratica sia saltato. C'è stato oggettivamente un modo di procedere che, sul terreno della minima sensibilità di carattere istituzionale, avrebbe determinato la capacità di riconoscere, al di là degli intendimenti, che peraltro sono legittimi nella dialettica parlamentare, parlamentare, che alcune questioni meritavano l'immediata sospensione della seduta e l'immediata convocazione della Giunta per il Regolamento per affrontare la questione. Questo è il dato di fatto, almeno dal mio punto di vista. Non si è determinato. Però la "sanzione" a quel che

Infatti il Presidente del Senato, per fare la proposta che ha fatto all'Aula, è dovuto partire da un presupposto, cioè che quelle votazioni sono irregolari, si sono effettuate in condizioni tali da determinarne l'irregolarità. Nel momento in cui il Presidente del Senato riconosce questo dato e prende atto di una situazione, seppure *ex post*, il problema che si pone sul terreno della cultura delle regole è se, ai sensi dell'articolo 118, la decisione assunta dal Presidente del Senato determini il riconoscimento di quell'«immediatamente» che è contenuto nell'articolo stesso, se cioè

riconosciuto dal nostro punto di vista con chiarezza quel che è accaduto, determinato il fatto che è stata riconosciuta l'irregolarità del voto, io credo che oggettivamente ci siano tutte le condizioni, per un comune senso di responsabilità istituzionale, per affrontare il tema: e il tema è, dal nostro punto di vista, riprendere le votazioni, rinnovare le votazioni, accantonare le questioni di cui si è discusso e si è parlato, rinviarle - come diceva il collega D'Alia - alla Giunta per il Regolamento e ripristinare - alla Giunta per il Regolamento e ripristinare all'interno dell'Aula del Senato un cammino condiviso rispetto alle regole che, credo, il senso di misura e di corretta interpretazione del Presidente del Senato cerca di ristabilire, tant'è che in sede di Conferenza dei Capigruppo tutti avevamo convenuto su questa impostazione, partendo da questo presupposto, che è un riconoscimento, cioè che le votazioni sono state irregolari. Prendiamone atto tutti e da questo presupposto cerchiamo di costruire un clima di responsabilità che ci faccia riprendere il dibattito e il confronto di merito su questioni così rilevanti e così importanti.

Non capisco questa discussione; non si può decidere *ex ante* di ripetere una votazione, ma dopo una discussione su una eventuale

chiarissima nell'abrogare alcune norme della precedente legge Moratti e nell'introdurre delle nuove regole, in particolare sul ruolo del professore aggregato. Quindi la volontà del legislatore emerge chiarissima dall'esame dei commi e dei vari dettagli. Peraltro, la questione che era stata risollevata oggi e che ha portato poi al momento di confusione era stata già al centro di una pregiudiziale, che era stata legittimamente presentata, credo dalla senatrice Bastico, ed era stata respinta dall'Assemblea. Il merito della questione lo discuteremo quando ci arriveremo in Aula o nelle sedi che si riterrà. Per quanto riguarda le votazioni, sinceramente adesso non voglio fare in questa sede una ricostruzione dettagliata dei fatti, ma è chiaro che la confusione in Aula è derivata dalle forti contestazioni provenienti dai banchi dell'opposizione per la questione di merito: quindi si chiedeva di non procedere nelle votazioni. Questo è un dato oggettivo che i colleghi non possono non riconoscere: si chiedeva a viva voce la sospensione della seduta e delle votazioni, quindi si è creata una condizione in cui il singolo senatore ha avuto grandi difficoltà nella normale comprensione delle proposte, delle votazioni, degli annunci e delle comunicazioni. Pertanto, c'è stata una contestazione di merito, che già le pregiudiziali avevano respinto; c'è stata una contestazione alla Presidenza che tutti abbiamo visto e che ha reso difficoltosa per i singoli parlamentari la comprensione delle indicazioni e dei richiami; non c'è stata nemmeno, per la concitazione dei momenti, una controprova. Credo peraltro che il senatore D'Alia abbia con correttezza rilevato che in quel momento c'era una maggioranza in Aula e dunque con la controprova o con altre richieste sarebbe stato facile riscontrare, come nelle votazioni precedenti, un orientamento favorevole al testo giunto dalla Camera. Concludo dicendo anche che la ripetizione del voto che il Presidente dispone sulla base del Regolamento e che ha numerosi precedenti non non solo deriva da una richiesta di tutti i Capigruppo avvenuta negli incontri, ma è stata avanzata per prima (lo devo dire con onestà e non posso essere smentito) dalla presidente Finocchiaro,

meno opinabile. Quindi, condivido la decisione del Presidente, quella che, aveva chiesto peraltro, la presidente Finocchiaro in presenza di tutti noi Capigruppo e che noi avevamo condiviso. Si Si possono cambiare le carte in tavola, ma io credo che ciò che aveva chiesto la presidente Finocchiaro, per la confusione che c'era stata in Aula, e ciò che comunque dispone il Presidente sia un atto di saggezza per consentire all'Assemblea di deliberare con responsabilità e in un clima dei nostri lavori Presidente, intervengo perché è doveroso che tutti coloro che sono stati parte di quella decisione

tutti siamo consapevoli che l'eccezionalità di questa vicenda (perché di questo si tratta) merita una puntualizzazione e una precisazione dei suoi contorni, perché la preoccupazione che il collega D'Alia ha manifestato mi appartiene pienamente. Se dovessimo uscire da questo caso anomalo (perché di questo si tratta), potremmo introdurci in una prassi che mette davvero a rischio la certezza dei lavori parlamentari.

però devo rendere testimonianza che lei correttamente ha riferito di aver assunto la decisione della ripetizione quando non c'era la consapevolezza di questa difformità delle proclamazioni, quindi al buio. Se questo non è titolo titolo di merito, è titolo certo che tutti abbiamo pienamente apprezzato. È altrettanto vero, con un principio sostanziale che però si lega poco alle forme parlamentari, che la maggioranza d'Aula era da un'altra parte, quindi quelle approvazioni sono nella sostanza il frutto della concitazione. Credo quindi sia giusto che ciò rimanga agli atti, perché non vi possono essere precedenti di questo tipo, determinati anche, voglio dirlo, da una forzatura

che dovrebbe sempre assistere i lavori parlamentari; invece, questo modo di intendere anche le appartenenze, questo clima da stadio, da tifoseria in cui si sta da una parte non ascoltando mai le altre parti ha determinato un incidente

Presidente, quando c'è una condizione di tumulto nell'Aula, il Presidente in esercizio sospende i lavori. Sono state assolutamente ineccepibili le considerazioni portate dal collega Li Gotti, il quale ha ricordato come la Presidente, di fronte alla sollecitazione per la sospensione dei nostri lavori, ha ripetutamente dimostrato, secondo la propria intenzione, di essere in piena padronanza dello svolgimento della seduta. Io invece sono del suo stesso avviso, cioè che quelle votazioni fossero irregolari: tanto questo è avvenuto che, nonostante il tumulto venisse accresciuto da un atteggiamento di alcuni senatori della maggioranza, i quali in modo tambureggiante invitavano la Presidente a proseguire, che io ho cercato di prendere la parola per fare una dichiarazione di voto su ciascuno degli emendamenti che venivano presentati, e questo era manifestamente impossibile perché, appunto, la Presidente aveva non la padronanza dell'andamento dei lavori, ma un desiderio quasi spasmodico di portare a conclusione la sua tesi, impedendo in questo modo a quei senatori che volevano chiedere la sospensione della seduta, chiedere di intervenire mentre proseguivano le votazioni, di poterlo fare. È evidente che quelle votazioni erano irregolari, però lei, signor Presidente, deve risolvere - e anch'io mi associo ad un esercizio di responsabilità che tutti cerchiamo di fornire in questo momento e che effettivamente, come ricordava il collega Pistorio, abbiamo

com'è possibile che si approvino qui delle norme che sono palesemente contraddittorie e tali da poter aprire la possibilità addirittura di un rinvio alle Camere

norme così palesemente contraddittorie, pur in presenza magari di una decisione interpretativa della Giunta per il Regolamento, non ottengano l'effetto di essere rimandate alle Camere dal Presidente della Repubblica, cosa che secondo me sarebbe la frittata conclusiva della senatrice Sbarbati).* Il primo problema è questo, e riguarda il rapporto tra il Governo e il Parlamento, poiché la materia è emersa in un modo così significativo. Il secondo problema riguarda quello che lei ha appena detto, cioè l'accantonamento

dell'attività dell'Aula, con la votazione di altri emendamenti. Se così avvenisse, signor Presidente, verrebbe meno proprio quello che lei richiamava, cioè l'immediatezza dell'annullamento del voto. Se lei adesso sospende e non annulla quel voto procedendo alla sua ripetizione, e passa ad altri

non faccia precedente, perché non sfugge ai colleghi, oggi della maggioranza o dell'opposizione che, se si stabilisce il principio in base al quale un emendamento dell'opposizione, accolto

dell'opposizione, approvato, possa poi dalla stessa maggioranza essere dichiarato invece decaduto, irregolare e respinto, se andassimo in una direzione del genere, creeremmo un precedente molto delicato. Per cui la mia sollecitazione è che su questi tre punti il Presidente proponga all'Assemblea una via d'uscita, auspicabilmente condivisa. Ripeto: in primo luogo, sul testo di questo provvedimento, in maniera tale che non ci ritroviamo domani ad accorgerci di aver approvato qualcosa che non poteva esserlo; secondo luogo, non procedendo adesso con la trattazione di altri articoli, così facendo venir meno l'immediatezza dell'eventuale correzione del voto che si sia dichiarato irregolare; in terzo luogo, stabilendo che non si forma qui un precedente, che in questo caso non avvantaggerebbe il Senato, ma una maggioranza che domani potrebbe lamentarsi di un precedente di questo genere.

la programmazione dei lavori in modo da tener conto della particolare delicatezza istituzionale e politica, così da non prolungare in maniera irresponsabile i nostri lavori. Le suggerirei di fare un *settlement* di queste questioni aperte, senza avventurarci nei guai. Le suggerisco di farlo adesso e di riconvocare la seduta - se necessario - tra un'ora, con l'intesa dei Capigruppo, e di proseguire

Senatore Rutelli, ho ascoltato tutti gli interventi e per ultimo il suo. Mi conforta sulla decisione che ho annunziato a inizio di seduta - e che confermo - il fatto che alcuni colleghi, sia di maggioranza che di opposizione, hanno avuto la bontà di ricordare come la mia decisione di rinnovare le votazioni fosse stata adottata, su richiesta dell'opposizione, su richiesta dell'opposizione, nella totale ignoranza degli episodi in ordine alla dichiarazione di approvazione o meno di alcuni emendamenti da parte del Vice Presidente di turno. Questo è stato riconosciuto, e ringrazio coloro i quali, partecipando alla informale Conferenza dei Capigruppo, erano presenti e hanno dato atto che la Presidenza del Senato, su richiesta dell'opposizione, aveva aderito dicendo che quelle votazioni, realizzate in un clima di conflittualità e di irregolarità,

la situazione di ingestibilità dell'Aula. Ciò, tra l'altro, confligge con quella che poteva essere - ed era stata sino a quel momento - la volontà palese e costante della maggioranza di respingere tutti gli emendamenti.

il senso dello Stato che lei mi ha riconosciuto, immeritatamente. Lungi da me l'idea, con le mie dichiarazioni e le mie scelte, di andare in questo senso. Lo faccio perché, quando avevo deciso di ripetere le votazioni, il suo Capogruppo, senatore Felice Belisario, era presente ed era d'accordo sulla ripetizione. Le posso assicurare che se questa decisione fosse stata adottata *a posteriori*, cioè quando la Presidenza avesse avuto notizia di questa anomalia, sicuramente la mia coscienza avrebbe avuto l'esigenza di una maggiore riflessione. Questo lo devo dire. La mia decisione, era stata assunta in buona fede, senza che nessuno dei presenti fosse al corrente di quello che era successo nella proclamazione degli emendamenti. Sulla decisione di rinnovare le votazioni, io mi sento, in piena coscienza, di fare una cosa giusta nel rispetto del Regolamento e anche della volontà dell'Aula, senatore Rutelli e colleghi senatori. Non vi è dubbio, secondo l'andamento dei lavori che da due giorni si prolungano, la volontà della maggioranza e la volontà dell'Aula è stata costante ed uniforme. Quindi, sono tanti i motivi che mi portano a dichiarare l'esigenza di annullare quelle votazioni e di ripeterle.

da parte della stessa presidente Finocchiaro, si è detto che quella richiesta era finalizzata a rispondere allo *speech* della presidente Mauro, ma che essa non risolveva *in nuce* il problema.

della ripetizione del voto mi sono pronunziato; su questo mi sono pronunziato. Si è poi affrontato anche un altro tema, come è stato accennato, ma, dal momento che è un problema di coordinamento e non un tema di sostanza,

Signor Presidente, il Governo, alla luce delle questioni di coordinamento sollevate dall'opposizione in merito ai reciproci rapporti fra i commi 4 e 5 dell'articolo 6 e l'articolo 29, si impegna a risolvere tali problemi in sede di conversione del decreto-legge di proroga termini che il Consiglio dei ministri approverà nella mattinata di domani.

innanzitutto mi consenta una replica assolutamente pacata al presidente Bricolo, che ha usato parole inaccettabili all'indirizzo del nostro Gruppo, ricordando a lei che noi non abbiamo speso neanche mezza parola

compiendo atti gravissimi. Signor Presidente, personalmente ho sempre tenuto e terrò un comportamento corretto e di stima nei confronti della presidente Mauro. Mi sono avvicinato a lei con il Regolamento in mano pronunziando esclusivamente le parole:

si voglia contestare la presunta esuberanza dell'atteggiamento dell'opposizione su una decisione, quella della presidente Mauro, che lei, signor Presidente,

Regolamento, che parla di irregolarità delle votazioni, cioè delle irregolarità di tutto ciò che avviene nell'emiciclo, di tutto ciò che viene

essere revocabili, ma bisogna procedere nell'immediatezza del fatto, non dopo che il fatto della decisione è stato cristallizzato nei verbali ed ha fatto il giro verbali ed ha fatto il giro dell'Italia, e non solo. Tutta Italia sa che quattro emendamenti sono stati approvati le cui votazioni lei, applicando una norma regolamentare che nulla c'entra con questa fattispecie secondo la nostra opinione, vuole annullare rinnovandole.

il comma 5 dell'articolo 6.

La Presidenza, in presenza anche di suoi colleghi di Gruppo, ha contattato la Presidenza del Consiglio per verificare se nel decreto milleproroghe si potesse già inserire questa correzione,

sta facendo - a questa argomentazione. Abbiamo tre norme di segno diverso tra di loro, di cui una può essere approvata. Vogliamo provare a tenerne due, in questo testo, per non calpestare il Regolamento e tutti i principi che sovrintendono al procedimento legislativo? L'unica soluzione plausibile, signor Presidente, è quella di accogliere l'emendamento 6.21, che sopprime il comma 5

allora ciò sarebbe molto grave, signor Presidente. La soluzione sta nella soppressione del comma 5 dell'articolo 6. Se lei farà votare a quest'Aula questo emendamento soppressivo, per poi metterci davanti ad una preclusione in quanto non è stato presentato l'emendamento soppressivo della norma abrogativa contenuta nell'articolo 29, saremmo in presenza di una arbitrarietà nell'arbitrarietà. Sono convinto che lei non voglia arrivare a questo punto. Siamo disponibili, come ha detto la presidente Finocchiaro, ad

dei suoi poteri e delle sue funzioni*,* che non possa apportare neanche mezza modifica ad una norma che è necessario modificare. Signor Presidente, premesso che non torniamo sull'applicazione dell'articolo 118 del Regolamento perché è una sua decisione, il dibattito è stato riaperto dalla dichiarazione dichiarazione del Ministro sulla seconda questione che riguarda i profili di ammissibilità di alcuni emendamenti. non riesco a comprendere la ragione per la quale si introduce - lo dico incautamente - il tema del decreto milleproroghe rispetto, ad una legge come correttamente ha detto lei che è ancora in fase di discussione e di approvazione in Parlamento, Parlamento, perché questo rischia di confermare la tesi che il collega Legnini sta sostenendo, cioè che c'è la necessità di correggere il testo per cui l'eventuale preclusione di emendamenti sarebbe un atto contrario all'articolo 97 del Regolamento. Farei allora finta di non aver ascoltato

perché o noi risolviamo la questione nell'ambito di questo procedimento legislativo oppure quell'emendamento deve essere messo in votazione. credo sia necessario che la Giunta si riunisca e affronti la questione. Ci sono anche precedenti a mia memoria che riguardano eventuali ordini del giorno interpretativi, di cui ha parlato anche il collega

in questo momento conoscenza del merito della questione, né ho la presunzione di affrontarla qui. Essa va affrontata in sede di Giunta per il Regolamento, che è il suo organo di consulenza per le questioni più complesse. Altrimenti, non ne usciamo, credo che il preannuncio di una modifica di un testo che ancora deve essere approvato sia una pezza che è peggio del buco. Sono del parere che di ciò non dovremmo obiettivamente tenere conto perché sembra

senatore Zanda,

ambedue consistenti. Vi è anzitutto un errore evidente, dalle conseguenze consistenti del Governo e della maggioranza alla Camera, al quale adesso il ministro Gelmini ha indicato una soluzione. Vi è poi una Presidenza, che eufemisticamente vorrei definire anomala, della Vice Presidente di turno che ha fatto proseguire in condizioni assolutamente impossibili la seduta,

soltanto che Governo e maggioranza accettassero un breve ritorno del provvedimento alla Camera dei deputati. Questa soluzione non viene accettata, né dal Governo, né dalla maggioranza, e ci troviamo quindi davanti a questa duplice decisione. Vi è anzitutto una decisione del Governo di presentare, se non ho capito male, un emendamento al prossimo emanando decreto milleproroghe, milleproroghe, che sarà certamente dichiarato inammissibile perché non si tratta di una proroga, quindi non si vede in che modo possa modificare un decreto milleproroghe. Ci troviamo poi davanti ad una

Finocchiaro e Legnini) sette voti in blocco. Ora, la considerazione politica, signor Presidente, è questa, e riguarda la Presidenza del Senato: vedo nella somma di queste due decisioni un modo per far giocare contro l'opposizione dei vizi e dei difetti che sono, viceversa, della maggioranza, del Governo e della Presidenza *pro tempore* del Senato di usare contro l'opposizione quelli che sono stati dei difetti della maggioranza e del Governo francamente, devo dirlo, mi sembra inaccettabile.

La mia decisione era stata assunta prima. La ringrazio, signor Presidente. In fondo l'intervento dell'onorevole Ministro va nella direzione, come è stato poc'anzi ricordato dal senatore Legnini e dal senatore Zanda, della bontà del voto con cui si è approvato l'emendamento 6.21. L'abrogazione

va fa altro che introdurre l'abrogazione del comma 11. Quindi, non sorgerebbe nessun contrasto se la modifica non venisse introdotta - è questo l'elemento di contraddizione - e poi venisse abrogato quel comma 11. Il paradosso è proprio questo: è stato proclamato

L'intervento di modifica solo su un emendamento significherebbe un passaggio velocissimo alla Camera, perché riguarderebbe soltanto questa norma, si tratterebbe proprio di poter fare qualcosa in ore. Invece, secondo quello che ha sostenuto e ha proposto il ministro Gelmini, dobbiamo portarci dietro una norma che è in conflitto con se stessa.

Sicché, ci troveremmo ora nella condizione per cui, secondo le indicazioni e le dichiarazioni del Ministro, andremmo a votare un emendamento che voi vorreste, ma che non potete votare. Noi vorremmo invece - ma a questo punto lo dobbiamo votare

l'emendamento soppressivo non venisse approvato, perché sarebbe meglio. Questo è un paradosso,

una serie di articoli che introducono le diverse modalità di voto dell'Assemblea, 113, 114, 115, 116 e 117, che prevedono le diverse modalità, e poi vi è - appunto - la norma di chiusura, che prevede la possibilità di reiterare una votazione irregolare, espressa in una delle qualunque modalità prescelte.

«Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni del Senato: se pronunziate, non si inseriscono nel processo verbale e nei resoconti della seduta». ai sensi dell'articolo 111 del Regolamento, è stato proclamato un voto, non sono ammesse neanche le proteste; se queste vengono pronunciate, non vanno neanche a verbale

L'*impasse* che si è creata stasera in quest'Aula non dipende, né dalla maggioranza, né dall'opposizione del Senato, ma certamente nessuno potrà non riconoscere che l'opposizione è stata seria e responsabile perché avrebbe potuto tacere; si sarebbe potuto procedere nella votazione nel silenzio più assoluto, non evidenziando come questo testo entri in profonda contraddizione. Se così fosse avvenuto, il provvedimento sarebbe tornato all'esame del Parlamento perché il Presidente della Repubblica

Non consentirò mai che qualcuno impedisca all'Aula di lavorare. Abbiamo parlato, parliamo da un'ora e mezza, se lei intende non lavorare non lavori. Per l'amor del Cielo! Noi abbiamo un impegno ed io intendo rispettare gli orari dell'Aula.

annullo le precedenti votazioni ed accantono l'emendamento 6.21, in maniera tale che non si possa pensare che da parte della Presidenza ci siano forzature. Le votazioni realizzate prima della mia Presidenza sono annullate e vanno ripetute. Possiamo però

Lei ne sta accantonando alcuni; credo siano tre. Quali sono quelli oggetto della precedente votazione annullata, in via di rinnovazione, che lei sottopone nuovamente all'Assemblea? Questa è la domanda.

Senatore Morando, stia tranquillo che stiamo operando in piena trasparenza.

grazie alla cortesia del Presidente, incalzato dalle domande del senatore Legnini, abbiamo appreso che in quest'Aula si sono fatte quindici votazioni nelle condizioni descritte; emendamenti votati, tre saranno accantonati. In conseguenza delle cose che sono state dette prima da me, dal senatore Legnini e dal senatore Zanda, volevo annunciare che il nostro Gruppo non parteciperà a nessuna delle votazioni che ritornano su decisioni che sono già state sottoposte all'Aula, come i verbali del Senato testimoniano.

in quest'Aula oggi non sia stato usato con la stessa logica e la stessa coerenza. Infatti, se avessimo adottato questo principio, oggi stesso, con la stessa logica, avremmo dovuto ripetere le votazioni in cui è stato accertato che il ministro Bondi aveva votato per un collega. Quando è stata sollevata l'obiezione su questo fatto, è stato detto che siccome la vicenda è venuta a conoscenza della Presidenza dell'Assemblea solo un'ora e mezza dopo, non si poteva più intervenire perché era venuta meno l'immediatezza.

quest'Aula aveva a portata di mano la possibilità di risolvere la questione e anche qualcuno della maggioranza lo ha fatto presente: si poteva accantonare la votazione sul primo emendamento relativo al comma 5. Non è stato fatto, a mio parere la votazione è andata come sappiamo e a questo punto, per risolvere il problema, bisognerebbe accettare il fatto che, essendo stato votato, il provvedimento deve tornare all'esame della Camera come hanno già detto molti altri colleghi. Non volete farlo, quindi ve ne assumete la responsabilità; noi non siamo d'accordo

di chiederle, apprezzate le circostanze, di togliere la seduta, anticipare la Giunta per il Regolamento e proseguire i nostri lavori domani. Forse sarebbe meglio, perché probabilmente anche sulle questioni poste la Giunta per il Regolamento potrà dire qualcosa in più;

che noi rappresentiamo il potere legislativo, questo mi pare evidente. Le leggi vengono formate ed approvate in questa sede. sede. Se noi rileviamo delle anomalie in questo disegno di legge e non lo modifichiamo in questa sede, ma diciamo che lo farà dopo il Governo, stiamo rinunciando alle nostre prerogative e ai nostri poteri.

ma, d'accordo con il Governo, diventa il braccio esecutivo del Governo. E siccome il Governo dice che questo disegno di legge non può essere rinviato alla Camera, allora voi non vi avvalete più delle vostre prerogative! Questa è una cosa che non si può tollerare, per cui se devo rimanere a lavorare qui, signor Presidente, e sentirmi bocciare tutti gli emendamenti che sono stati presentati, io mi allontano da quest'Aula e non ci torno più.

Solo in punta di Costituzione, senatore D'Ambrosio: è vero che la separazione dei poteri, visto il potere dove lei si trovava, fino a poco tempo fa, è cosa che conosce bene. Ma detto questo, lei dovrebbe sapere che il regime parlamentare si fonda sulla comunicazione del potere legislativo e del potere esecutivo, perché quello a cui lei si riferisce è il sistema presidenziale, che a me piacerebbe tanto avere nel nostro Paese, ma che invece non c'è. Questo Parlamento, questa maggioranza che comunica con il suo Governo, ha preso semplicemente atto di una dichiarazione del Governo e sulla base di questa si regola e regola le sue prerogative. Lei potrà non essere d'accordo, ma non può pensare di trattare i poteri dello Stato non secondo la Costituzione e gli schemi formali, ma secondo la sua fantasia. Si studi cosa è un regime parlamentare prima di dire certe cose in un'Aula del Parlamento.

di un testo complesso. L'emendamento 6.41, che ha una sua importanza non solo terminologica, mette più chiaramente in luce l'oggetto che si vuole tutelare.

di correggere, per una volta almeno, se possibile, un termine sbagliato, in questo contesto che è sbagliato anche per altri. Questo emendamento ha un suo valore e vi prego di appoggiarlo.

questo emendamento si colloca in un contesto che è segnato in profondità dalla sottovalutazione del ruolo del senato accademico e dalla sopravvalutazione volontaristica del ruolo del consiglio d'amministrazione. Noi riteniamo che questa logica contenga un profondo errore di impostazione, che questa legge vuole a tutti i costi compiere e che noi, invece, cerchiamo di limitare. Il senato accademico, con tutti i suoi difetti virtuali, è l'espressione della comunità scientifica ed è composto da persone che hanno, se non altro, attraversato i compiti della formazione e della ricerca e che hanno idea di quali siano i compiti della comunità scientifica. Il consiglio di amministrazione è, per sua definizione, un organo che risponde a una filosofia di natura diversa, incardinato sui temi della gestione economica e delle ragioni di spesa. Quindi, sottrarre la guida dell'università al senato accademico comporta l'enfatizzazione di una filosofia di natura aziendalsitica, che è in perfetto accordo con la filosofia dominante in questa maggioranza, che vede nelle ragioni di azienda il "termine fisso d'eterno consiglio". Però, di fronte a questo, proprio per questo, nei limiti del possibile dell'attività emendativa, noi compiamo lo sforzo di ridare, potestà significative al senato accademico. Questo emendamento si colloca proprio dentro questa logica.

ha un suo valore. Tutto questo testo, infatti, è stato classificato, nella comunicazione pubblica, come la riforma della *governance* dell'università. Questo è stato lo *slogan* privilegiato del Governo.

che una legge delega, che dovrebbe in qualche modo demandare queste norme agli statuti dei singoli atenei, delle singole università, vada ad interessarsi

un emendamento che evidenziava la necessità del parere delle Commissioni parlamentari. In questa sede più volte abbiamo sottolineato come viene svalorizzato il ruolo del Parlamento, e in questo caso delle Commissioni parlamentari, rispetto a temi

può apparire come un emendamento che, aggiungendo una bardatura governativa ad una libera attività universitaria, da un certo punto di vista potrebbe apparire sommamente criticabile. In realtà, più di quanto potesse la lucidità mia in questo momento, la collega Bastico ha trovato le parole giuste per dargli una motivazione, cioè che il ricorso all'interesse delle Commissioni parlamentari può essere uno strumento di stimolo, utile anche nel colloquio interno tra commissioni parlamentari e università. Visto l'emendamento in questa luce, l'autonomia universitaria non ne risulta lesionata, ma anzi è in un certo senso irrobustita dal dialogo con il livello istituzionale. Trovo quindi che il suggerimento della collega Bastico sia straordinariamente efficace.